Onorevoli colleghi, prima di proseguire nell'esame del bilancio interno, desidero comunicare che oggi, alle ore 14,30 circa, si è verificata un'interruzione nell'alimentazione elettrica da parte dell'azienda fornitrice. Ciò è accaduto anche in altre zone della città. Secondo i previsti tempi tecnici, sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni, che hanno consentito l'alimentazione dell'illuminazione di tutti i palazzi e della forza motrice nei palazzi centrali. Tali gruppi elettrogeni sono rimasti in attività fino al ristabilimento delle condizioni di esercizio da parte dell'ente fornitore, avvenuto circa un'ora dopo l'interruzione. Sono inoltre stati disattivati, in via cautelativa, gli ascensori in alcuni dei palazzi centrali. Sono attualmente in corso ulteriori verifiche di funzionalità, ma allo stato non risultano particolari problematiche in essere. **Seguito della discussione L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei Documenti VIII, n. 3 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2008) e VIII, n. 4 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2009).

la proposta di accorpamento dei Servizi studi della Camera e del Senato e il problema del riconoscimento della figura professionale dei collaboratori parlamentari. Per quanto riguarda la prima

di una dimensione naturale del bicameralismo, anche se il Parlamento nel suo insieme invece riuscire ad esprimere anche una unitarietà di funzioni: l'ambito dei Servizi studi appartiene più al terreno dell'unitarietà che non a quello della concorrenzialità. Per generale ammissione, i Servizi studi di Camera e Senato sono degli organi di straordinaria validità, composti da persone di grande preparazione e di grande competenza professionale. Nasce il dubbio dell'utilità di tale separazione, giacché

quella di disporre di schede di accompagnamento per ogni provvedimento in forma tempestiva, in modo tale da permettere ai Gruppi parlamentari di usufruire di tale vantaggio. Rilevo, *en passant*, che nell'esperienza accumulata di recente ho registrato che non sempre tutti i provvedimenti sono stati accompagnati da schede informative e non sempre la tempestività è stata garantita. È capitato talvolta che i Gruppi parlamentari abbiano dovuto affrontare discussioni urgenti su argomenti molto ricchi e pieni di problematiche disciplinari interne ardue in tempi strettissimi, con una certa difficoltà di documentazione autoctona.

però veramente insopportabile il brusìo che c'è in questo momento nell'Aula, anche perché si discute di cose che vi riguardano direttamente, che concernono la vostra funzione e i vostri compiti. Prego, collega Pardi,

cui ci fosse l'intenzione di progettare un trasferimento simile a entità esterne, penso che dovremmo meditare a lungo e con profonda serietà su questo che sarebbe a nostro avviso un errore basilare, per un motivo elementare: la conoscenza della materia legislativa dall'interno e l'acquisizione degli elementi interpretativi sui provvedimenti devono poter essere fondate sulla certezza dell'imparzialità degli estensori dei pareri, delle opinioni e delle indicazioni bibliografiche. Non si può neanche per un secondo sospettare che la materia offerta ai Gruppi parlamentari dai Servizi studi sia immaginata,

ravviso due elementi: uno triviale e l'altro di senso. L'elemento triviale è che non si capisce perché si debba spendere per andare a richiedere tali servizi all'esterno quando c'è già una struttura ottima all'interno che li garantisce. L'elemento di senso è quello che accennavo prima, e cioè il fatto che la garanzia dell'imparzialità può essere richiesta e fortemente voluta da parte di una struttura interna, mentre non c'è nessuna garanzia che sia data da una struttura esterna. Stando così le cose, noi chiediamo che ci sia un rafforzamento del Servizio studi nell'ottica di una maggiore connessione tra il Servizio stesso e le segreterie delle Commissioni permanenti, speciali, bicamerali, di inchiesta, nonché dell'Assemblea, con l'obiettivo di fornire tempestivamente ai senatori schede di lettura su ogni singolo Chiediamo inoltre che si promuova la progressiva unificazione del Servizio studi del Senato della Repubblica con quello della Camera dei deputati, indirizzandosi verso la costituzione di una sorta di Servizio studi del Parlamento della Repubblica nel suo insieme, con l'obiettivo di una maggiore efficienza ed efficacia nel rispetto dell'economicità dei lavori e del risparmio delle risorse. Chiediamo infine che si valuti la possibilità di integrare le preziosissime schede di lettura elaborate dal Servizio studi con una breve rassegna stampa tematica riferita al provvedimento in oggetto, contenente gli articoli di rilevanza dottrinaria ed altamente specialistica apparsi sulle principali riviste giuridiche, sia cartacee che *on line*, nonché quelli pubblicati dalle più importanti testate giornalistiche nazionali.

il problema annoso e per un certo aspetto anche drammatico dei collaboratori parlamentari. Negli ultimi tempi, sono state fatte varie indagini

Prendiamo atto del fatto che questa mossa, che aveva una perfetta giustificazione, in realtà non ha raggiunto il suo effetto. Allo stato attuale, alcuni sondaggi molto significativi attesterebbero che circa il 62 per cento dei collaboratori della Camera è in nero, e non è improbabile che questo accada anche al Senato. Lasciamo in sospeso la cifra: non conta la cifra, ma l'esistenza di un fenomeno che per definizione

cancellare il problema del lavoro nero nella società, ma è veramente pazzesco che non si sia in grado di farlo nemmeno all'interno delle Assemblee elettive. Questo impegno deve Questo impegno deve diventare primario. Non si può accettare la soluzione intervenuta dopo il tentativo operato dal presidente Bertinotti nella legislatura precedente precedente e che si è realizzata attraverso il trucco di far passare i propri collaboratori come ospiti temporanei:

evidentemente pone un problema di ordine sociale all'interno della nostra Camera.

è l'elemento di senso fondamentale - nelle condizioni perfette, dovrebbe avere con il parlamentare un rapporto personale, saldato dalla fiducia reciproca e basato anche su una fiducia di natura disciplinare, di conoscenza, di approfondimento comune, sulla capacità di indagine sui nuovi problemi aperti e quindi anche una certa tendenza alla co-ricerca, all'interpretazione dei fatti nuovi che si presentano. Questo tipo di rapporto si può fondare soltanto su una profonda sincerità nei rapporti personali e sulla solidità dei rapporti istituzionali. Se si entra nell'ordine di idee che il collaboratore parlamentare è un qualsiasi co.co.co. che viene pescato a turno dall'esterno in modo fortunoso, casuale e probabilmente anche ciclicamente disordinato

essendo un lavoro serio, *in progress*, sull'attività legislativa deve essere fondato su una grande saldezza, e quindi impoverisce la natura stessa del lavoro che deve essere svolto.

problema ad un'autorità esterna, ci si libera della responsabilità personale e questo è un aspetto che, secondo me, il singolo parlamentare, prima che la

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di estendere ai collaboratori dei Senatori il regime già previsto per i collaboratori dei componenti del Consiglio di presidenza e dei Presidenti di Commissione, ossia il versamento diretto da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica, dei compensi stabiliti in favore dei collaboratori stessi.

più da santo inquisitore che da collega senatore. Lo ha bocciato interamente, distruggendolo per mancanza di chiarezza, trasparenza e quant'altro. Io francamente inizio il mio intervento per dissentire da questa interpretazione, perché ritengo che quest'anno il bilancio del Senato, rispetto agli anni precedenti, sia più chiaro e trasparente,

di un obiettivo di sempre maggiore chiarezza e trasparenza nella comunicazione dei nostri documenti di bilancio, e soprattutto dell'attività amministrativa di cui essi sono espressione». Facendo seguito a seguito a questo intendimento del Collegio dei Questori, intendo proporre nuovamente qualche mia vecchia proposta, che chiedo sia esaminata con l'attenzione che riterranno opportuno prestarvi. bilancio interno del Senato quest'anno, per la prima volta (almeno per quanto mi riguarda nella mia esperienza triennale di senatore), sono stati messi a disposizione 15 giorni prima e, di conseguenza, tutti ne hanno avuto contezza e hanno potuto fare le proprie osservazioni. La prima questione che pongo è sempre quella del *quorum*. A mio avviso, un documento così significativo e importante avrebbe bisogno di un *quorum* sia per la discussione che, a maggior ragione, per l'approvazione. Non vorrei essere confuso col cognome sbagliato del senatore facendo una predica anch'io, però francamente mi sembra un elemento da valutare con la dovuta attenzione.

che raccolga in un testo unico integrato i numerosi provvedimenti, che oggi regolano la materia, con indicazioni normative non sempre chiare e coerenti tra loro e che suscitano qualche perplessità interpretativa sulla natura di tali fondi e sulle concrete modalità applicative». E ancora, a pagina 20, è detto: «È peraltro noto che la spesa obbligatoria, pagata a ruolo sulla base di disposizioni contenute direttamente nei regolamenti interni o in specifiche deliberazioni dello stesso Consiglio di Presidenza, è per sua natura non solo difficilmente comprimibile, ma rappresenta anche il fattore più rilevante di crescita della spesa complessivamente considerata». Ecco allora la mia seconda proposta: affrettare affrettare questo lavoro di riordino di tutte le disposizioni contenute nelle delibere assunte dal Collegio dei Questori nelle precedenti legislature e di quelle adottate dai vari Consigli di Presidenza che si sono succeduti,

si è aumentato notevolmente il *deficit* pubblico, fino a farlo diventare, negli anni '90, incontrollabile. Ecco allora che in quell'epoca storica era facile adottare nei Consigli di Presidenza o nei Collegi dei Questori, senza alcuna critica a chi a suo tempo ne ha fatto parte, una serie di deliberazioni che hanno costituito dei *benefit*, come io li ho definiti. Qualcuno preferisce chiamarli diritti acquisiti, ma io francamente li chiamerei piuttosto privilegi ingiustificati. Mi riferisco, ad esempio, a quelli - e vado a toccare un aspetto dell'ordine del giorno G5

al Consiglio di Presidenza, ai senatori Questori e Segretari e ai Presidenti di Commissione. Il capitolo delle spese relative al personale addetto

che probabilmente in altri momenti storici di particolare disponibilità finanziaria era forse anche possibile concedere appartamenti o uffici di rappresentanza a un numero notevole di componenti di questa Camera e, in particolare, a

avuto l'onore di entrare a far parte del Parlamento io, come del resto la maggior parte dei miei colleghi - svolgere interventi contro i cosiddetti privilegi dei parlamentari, per la riduzione di ogni qualsivoglia beneficio (erogazione, pagamento e rimborso) rivolto ad essi o a coloro che li aiutano a svolgere il loro compito. Nessuno può sapere se questi interventi sono fatti sapendo che tanto poi la maggior parte degli altri colleghi respingerà queste proposte oppure se sono fatti con sincerità: davvero questo non lo possiamo sapere. Possiamo sapere, però, che ciascuno di noi è libero di restituire quello che vuole della propria indennità o emolumenti (o comunque vengano chiamati): e non mi risulta che ci sia un grande affollamento presso l'apposito

quando parliamo delle spese del Senato (bilancio interno e compensi dei senatori) credo che innanzi tutto dovremmo sapere di cosa parliamo. Il bilancio parla di 532.158.987 euro: si tratta di

Dobbiamo farlo con questi 532 milioni e credo che dovremmo farlo con qualunque somma che come Parlamento e come Senato ci troviamo ad amministrare quando parliamo del bilancio e delle spese dello Stato. Oggi, però, parliamo di questa frazione: si tratta appunto di 532 milioni, più o meno 74 centesimi al mese per ogni italiano. Sarebbe questo, dunque, il risparmio che si realizzerebbe nell'ipotesi che di fatto sta dietro a molte proposte, che non dico certo vengano da quest'Aula, ma che si ventilano su

perché la pensione ai dipendenti dovremmo comunque pagarla: e si tratta di 82,5 milioni di euro all'anno. Quanto alle altre spese per il personale, che ammontano a 165 milioni, sarebbe davvero curioso troncarle da un giorno all'altro in un Paese che non ha mai licenziato un dipendente per il solo fatto che non ce n'è più necessità: si tratterebbe piuttosto di affidarli ad una chissà quale altra pubblica amministrazione, la professionalità dei dipendenti del Senato è in gran parte altissima e, peraltro, difficilmente impiegabile in altri campi, per cui si tratterebbe di un processo lungo, per cui si tratterebbe di un processo lungo, che richiederebbe parecchi anni. Di quei 165 milioni, almeno 40 si può calcolare che siano una partita di giro, se non per il Senato,

Quanto ai 48,8 milioni indicati nel bilancio per l'indennità parlamentare, ben 29 tornano al Senato in termini di contributi vari per il vitalizio o l'assistenza o allo Stato come imposte.

l'eventuale soppressione istantanea del Senato non farebbe risparmiare 532 milioni, ma solo 171 e altri 165 nel momento in cui si fossero proficuamente collocati altrove i 1.029 dipendenti (tanti risultano

vedovi che, all'età che verosimilmente hanno, difficilmente troverebbero un lavoro. In altri termini, già oggi, l'intera struttura del Senato non costa 532 milioni, ma non più di 440, dei quali una parte non irrilevante torna subito allo Stato in termini di IVA che il Senato paga su acquisti e forniture. Abbiamo, pertanto, un totale di 61 centesimi al mese per ogni italiano.

I rimborsi spese non sono delle retribuzioni; pertanto, la parola emolumenti comprende impropriamente in questo bilancio cose che emolumenti non sono: si tratta sicuramente di un costo sostenuto dal Senato, ma non sono emolumenti perché comprendono, infatti, le spese di viaggio

informatica, la diaria per il soggiorno a Roma (qualunque lavoratore dipendente si vede rimborsare le spese sostenute per raggiungere e soggiornare in una sede lontana da casa) e il necessario per soggiornare e pagarsi i pasti presso il Senato, o altrove, quando il ristorante del Senato è chiuso, per circa 20 giorni. Chi soggiorna a Roma meno di 20 giorni al mese indubbiamente può realizzare una qualche forma di risparmio da questo

61 milioni comprendono anche il contributo di supporto, una somma che non è esclusivamente destinata al compenso dei collaboratori, ma deve servire per tutte le altre spese inerenti la funzione del parlamentare, com'è indicato specificamente nel bilancio.

Non si tratta di lusso, ma di spese che uno evidentemente non affronterebbe se non fosse parlamentare e facesse un'altra attività. Questa somma viene generalmente definita "contributo portaborse". È interessante notare come in un Paese che definisce, per esempio, operatore scolastico colui che fa le pulizie in una scuola - cito questa nobile mansione, che ho l'orgoglio di avere praticato, solo a titolo di esempio; per cui, sia chiaro che ogni lavoro è pienamente rispettabile

Facciamo un piccolo ragionamento. Supponiamo di usare tutta la somma destinata a supportare nell'insieme l'attività parlamentare per pagare una sola persona. senza contare che poi dovremo pagare il consulente del lavoro che ci dirà come e quando svolgere i vari adempimenti, avremo una somma tre volte tre volte e mezzo inferiore, cioè una somma pari alla media del costo per ogni dipendente del Senato divisa per 3,5. Evidentemente, non è

ha un'indennità netta di circa 4.400 euro al mese. Nel gennaio 1990, chi fosse stato nella stessa situazione e con gli stessi oneri di oggi, avrebbe preso una somma in lire equivalente a 6.533 euro di oggi. Quindi, si è passati dai 6.533 euro del gennaio 1990 ai 4.349 euro del gennaio 2010, che è l'anno di cui ci occuperemo ben presto. Se poi ci si trova nella situazione di esercitare anche un altro privilegio (che è stato abolito e che viene per l'ultima volta esercitato in

va sempre contrapposta ai 6.533 euro del 1990, epoca nella quale, con vari meccanismi che sarebbe lungo spiegare, in pratica il riscatto lo si pagava sì, ma talmente più in là nel tempo che

Detto questo, si tratta di stabilire se queste somme siano adeguate, troppe o troppo poche: di sicuro, rispetto al passato, sono inferiori. Il giudizio, poi, va stabilito su una valutazione precisa perché, alla fine, abbiamo un costo - quello riferito alle indennità - pari a circa tre centesimi al mese per ogni contribuente.

la politica dell'Unione europea per l'adempimento degli obblighi che l'Unione europea ha scelto di assumersi rispetto al Trattato di Kyoto sulla politica ambientale e delle emissioni. Su questo si è già molto dibattuto in quest'Aula e spero che se ne parlerà ancora. 181 o 182 miliardi nel corso di 10 anni. Con questi si fa funzionare il Senato per 340 anni nel suo insieme e si pagano le indennità ai senatori per 9.000 anni. Certamente credo che una decisione oculata al riguardo valga la somma che si spende per il funzionamento di questa struttura. C'è chi, o per scarsa conoscenza dei numeri o per altri motivi o perché pensa davvero di non valere questa somma oppure per altri motivi che ho citato prima, continua a dire che bisogna ridurre, tagliare e così via. Ricordo che abbiamo l'impegno di non aumentare in termini nominali, dunque ridurre in termini reali alcuno emolumento o retribuzione o competenza ai senatori fino alla fine della legislatura, per cui anche di questo credo che andrebbe tenuto conto. Alcuni dei colleghi colleghi dell'Italia dei Valori hanno attaccato pesantemente il bilancio del Senato, parlando addirittura di poca trasparenza.

Signor Presidente, senatori Questori, colleghi, prendo lo spunto da un breve ordine del giorno che avrei dovuto illustrare questa mattina e che metto subito da parte anche per rassicurare il la trasparenza la chiediamo per noi e per tutti. L'ordine del giorno ha per oggetto un problema specifico, ossia la sistemazione dell'area di parcheggio intorno al Palazzo del Senato. Voglio essere molto breve in questo ma credo che vadano coniugate le esigenze dei cittadini residenti in quest'area, sempre per non far sì che il distacco tra i cittadini e il Palazzo aumenti, e le esigenze

Vi è una seconda questione, signori Questori, che credo vada assolutamente sistemata ed è la riserva di posti per la Presidenza del Senato

senza creare ulteriori privilegi. Non ne faccio una questione pregiudiziale, ma mi affido al vostro buon senso e credo che nel giro di poco tempo tale questione possa essere risolta. Ma il mio discorso, sollecitato da Malan e da altri colleghi questa mattina, credo vada assolutamente allargato. Ho ascoltato con soddisfazione, signor Presidente, l'annuncio della Presidenza di voler sollecitare i Gruppi

Siamo stati corretti, istituzionalmente rispettosi delle decisioni, ma adesso siamo arrivati al punto che in breve tempo anche il nostro Gruppo dovrà assolutamente essere rappresentato,

Come pure, in parziale dissenso con il mio Gruppo, vorrei dire in maniera molto chiara che pretendo da voi, dai Questori e dal Consiglio di Presidenza che finalmente venga salvaguardata la dignità del parlamentare. Siamo ormai stufi di essere attaccati sulla stampa da gente poco informata. Alcuni Gruppi si buttano a pesce nella marmellata, utilizzando e sfruttando notizie non vere

Una cosa è l'etica e la morale, di cui adesso parlerò, un'altra utilizzare, anche nel discorso che stiamo facendo questa sera, le cifre sentite da Malan.

senza vergognarsi. Ecco la trasmissione dei dati all'esterno: colloquiare con l'esterno senza assolutamente avere paura.

perché ognuno qui si circonda di rendite.

Vi pare che i Gruppi non debbano farlo? Credo che sia corretto che tutto ciò rientri in un complesso organizzativo generale che vada a ridare regole certe,

furbi; vanno innanzitutto previste anche nuove forme di assunzione, ma soprattutto va bandito il fenomeno del personale in prestito,

apprezzo l'impegno e lo sforzo di razionalizzazione del bilancio del Senato, che continua anno dopo anno, al fine del contenimento dei costi e dell'accrescimento dell'efficienza della nostra organizzazione. Il documento di bilancio che ci viene presentato per il 2009 è sempre più analitico e leggibile, e anche di questo mi compiaccio con i senatori Questori e con i Servizi competenti dell'Amministrazione. Ulteriori analisi e lo spacchettamento di diverse categorie di spesa sarebbero utili per meglio far comprendere anche all'esterno qual è il costo effettivo al netto delle imposte della funzione parlamentare, come ha sottolineato or ora il senatore Malan. Nella sostanza, il bilancio di previsione per il 2009 prevede la stabilizzazione della spesa complessiva a 594 milioni di euro, e questo è un obiettivo apprezzabile anche per l'immagine che il Senato proietta all'esterno. Se si esamina tuttavia la composizione della spesa, si evince che detta stabilizzazione è resa possibile essenzialmente, da un lato, dalla riduzione delle competenze dei senatori e dei contributi ai Gruppi parlamentari dall'altro, dalla riduzione della spesa in conto capitale, mentre continua a lievitare, anche se percentualmente di poco, la spesa per il personale di ruolo e a contratto del Senato, Senato, che rappresenta la percentuale evidentemente più importante di tutta la spesa corrente del Senato. Ciò avviene nonostante una riduzione significativa delle indennità di funzione e di risultato. Non basta quindi fissare l'obiettivo di tenere il personale al di sotto di 1.000 unità; la riduzione della spesa corrente richiede una riduzione dell'organico effettivo del Senato e una revisione dell'articolazione amministrativa del Senato stesso, di cui non c'è traccia nel bilancio che ci viene presentato. A questo riguardo mi riservo di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno G1, se necessario. Dichiaro inoltre di essere tendenzialmente contrario, almeno per quest'anno, a nuove spese e a nuovi strumenti e servizi resi ai senatori e alle Commissioni.

la mia personale soddisfazione, in quanto il dibattito sul bilancio interno rappresenta, come sappiamo, un'occasione di confronto di idee, di opinioni, ma anche e soprattutto un momento di concretizzazione di esigenze operative, di cui i senatori Questori potranno e dovranno tener conto nello svolgimento del proprio mandato amministrativo. Questa replica sarà svolta da me e dal collega Franco Paolo,

fare a meno di rispondere dettagliatamente a una serie di considerazioni che sono emerse durante il dibattito che c'è stato, augurandomi di poter dare al riguardo una risposta che risulti soddisfacente. Avverto l'esigenza di rispondere puntualmente all'intervento del collega Pedica, che voglio rassicurare anzitutto circa la preoccupazione da lui espressa sul vuoto esistenziale che ravvisa nel documento di bilancio. In realtà, il bilancio che i senatori Questori e il Consiglio di Presidenza sottopongono oggi all'Aula è in piena sintonia con lo sforzo generale di risanare la finanza pubblica e di riqualificare la spesa, offrendo un esempio di buon governo, ma soprattutto di rigorosa amministrazione. Vogliamo assicurare che gli impegni assunti per il 2009 sono concreti e vanno esattamente in questa direzione. Ribadiamo che le risorse allocate nelle poste di spesa sono la sommatoria complessiva degli impegni derivanti dai vincoli regolamentari e contrattuali vigenti, degli impegni residui registrati a consuntivo 2008 e del fabbisogno aggiuntivo stimato per garantire le ordinarie esigenze di funzionamento e di funzionalità dell'Istituzione, secondo un chiaro criterio di programmazione della spesa. il Collegio ha già da tempo adottato una metodologia di monitoraggio e di controllo della spesa che consenta, *ex ante*, la verifica puntuale del fabbisogno dell'amministrazione (fornendo degli indirizzi sulle linee guida nell'ambito del procedimento di gara) e, *ex post*, monitorando ogni singola spesa al fine di una verifica puntuale del rispetto dei requisiti previsti in contratto, in termini sia di livello dei servizi erogati che di costi. L'impegno del Senato è tangibile e verificabile sia sul versante delle entrate che su quello delle spese. Sul versante delle entrate, mi permetto di evidenziare la previsione dei contributi previdenziali aggiuntivi da senatori ed ex senatori a titolo di riscatto del triennio di completamento della XV legislatura, nella misura di circa 1 milione di euro; la previsione di ben 1,8 milioni euro di entrate aggiuntive da parte del personale per effetto dell'incremento a carattere permanente dei contributi previdenziali (che sono passati dall'8,8 al 9,7 per cento delle retribuzioni) e per effetto anche del contributo dello 0,75 per cento a carico dei trattamenti pensionistici diretti. Ci troviamo di fronte a una vera e propria diretta partecipazione di senatori e dipendenti alla formazione delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio del Senato, che naturalmente ci metteranno nella condizione di chiedere al bilancio dello Stato il trasferimento di minori risorse finanziarie. Sul versante della spesa, vogliamo sottolineare in particolare la flessione della spesa obbligatoria, che rappresenta la parte preponderante della spesa complessiva, nella misura complessiva dell'1,30 Inoltre, nella relazione di accompagnamento al bilancio abbiamo voluto riprendere una suggestione avanzata dal collega Baldassarri nel corso del dibattito sul bilancio interno in Aula lo scorso anno, riconsiderando la spesa obbligatoria secondo un criterio di aggregazione che differenzia la spesa finalizzata all'attività corrente da quella destinata ai trattamenti In tale chiave di lettura, gli interventi di controllo e di contenimento sul trattamento dei senatori e del personale dipendente hanno consentito addirittura una riduzione della spesa complessiva nell'ordine del 3,1 per cento. Per il trattamento previdenziale dei pensionati e dei vitalizi invece, che tra l'altro rappresenta quasi un terzo della manovra di bilancio, non possiamo che registrare gli effetti di incremento, pari al 3,51 per cento, determinati in buona parte dalla crescita del numero degli aventi diritti all'assegno vitalizio e dai nuovi collocamenti a riposo del personale dipendente ai quali si è prima accennato. Quanto alle altre spese destinate essenzialmente al funzionamento del Senato e, in particolare, ai servizi, ai lavori e alle forniture, che rappresentano un modesto 14 per cento della manovra complessiva, i dati sono di per sé eloquenti: l'abbattimento di circa 9,5 milioni di euro rispetto alle analoghe previsioni del 2008 con una flessione del 10,17 per cento è la diretta espressione della rigorosa valutazione del fabbisogno e dell'attenzione posta dai senatori Questori al risparmio. Ci riferiamo, in particolare, alle procedure di gara già concluse, che hanno consentito di trasferirne gli effetti positivi alla manovra di bilancio al vostro esame e a quelle calendarizzate per questo anno e illustrate ampiamente nella nota illustrativa che accompagna l'allegato n. 2, sez. *b)*, del bilancio stesso, in esito alle quali ci attendiamo risparmi anche più significativi rispetto alle previsioni. Rispondendo alle questioni particolari sollevate dal collega Pedica in materia di contratti in essere per forniture e servizi, desidero ricordare che nella tabella dell'allegato n. 2, appena richiamata, vengono elencati, pur nel doveroso anonimato dei soggetti destinatari, tutti i rapporti contrattuali vigenti classificati per tipologia dell'oggetto (locazioni, forniture, servizi eccetera), e indicando per ognuno di essi, da una parte l'incidenza in termini finanziari sul bilancio corrente, dall'altra la data di scadenza. La stessa nota illustrativa, che quest'anno abbiamo voluto predisporre a corredo dei dati schematici, è in grado di offrire con chiarezza ulteriori elementi di comprensione che, siamo sicuri, potranno soddisfare le richieste di carattere generale poste dall'intervento del collega. Entrando nello specifico, occorre tenere distinte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia comunitaria da quelle d'importo inferiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, il Senato della Repubblica indice procedure di gara aperte (precedentemente denominata asta pubblica) o ristrette (precedentemente denominata a licitazione privata), da giudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Ai sensi della normativa vigente sono assoggettati a pubblicità legale (vale a dire pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali europea e nazionale, oltre a quattro quotidiani e sito Internet dell'amministrazione) il bando di gara e l'avviso sui risultati della procedura. Gli atti intermedi della procedura sono accessibili ai sensi della legge n. Con riguardo ai capitolati, essi di norma non sono pubblicati sul sito Internet del Senato per prevalenti ragioni di riservatezza dell'istituzione parlamentare, come consentito dall'ordinamento di settore.

Da alcuni anni i senatori Questori non sono nominati componenti delle Commissioni aggiudicatrici. Sia i membri interni che gli esperti esterni indicati dai senatori Questori sono designati secondo criteri di alternanza. Il Collegio, al fine di uniformarsi a quanto prescritto dal codice degli appalti pubblici, ha deciso - in accordo con l'amministrazione - di proporre al Consiglio di Presidenza che venga istituita la figura del responsabile del procedimento di gara.

parità di trattamento e trasparenza. In ogni caso, a partire dal 2007, secondo l'indirizzo del Consiglio di Presidenza, tutti i principali servizi che fanno capo all'amministrazione del Senato sono stati accorpati in *global* o *multiservice*, secondo le norme europee. Quanto all'albo dei fornitori, l'amministrazione fin dal febbraio 2008 ha proposto uno schema di regolamento utile ad allineare detto strumento alle previsioni del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità. Nelle more, le iscrizioni all'albo sono sospese. Voglio in proposito ricordare che, a distanza di due anni dall'entrata in vigore dell'attuale regolamento di contabilità, la Presidenza e i senatori Questori hanno avvertito l'esigenza di procedere al monitoraggio sul concreto funzionamento della nuova disciplina, al fine di procedere a quegli adeguamenti che si dovessero rivelare necessari per conseguire obiettivi di semplificazione, maggiore trasparenza e razionalizzazione delle procedure amministrative. Per quanto riguarda la notizia sulla revoca del bando di gara edile-impiantistica, essa è stata chiesta dai senatori Questori con nota giugno 2009, in ragione di nuove esigenze di carattere prioritario e strategico, vale a dire quelle di una maggiore efficienza dei servizi legata ad un contenimento dei costi, nonché alle strategie in materia di risparmio energetico, e considerate

dell'uomo del 28 aprile scorso, che ha affermato la validità in linea di principio del sistema della cosiddetta giustizia domestica. Per quanto riguarda la questione della ristorazione, va precisato che la ditta "La Cascina" non è più presente in Senato sin dal 2006. In ogni caso non gestiva affatto in monopolio tutti i servizi di ristorazione del Senato, bensì solamente la caffetteria del personale e quella dei senatori. Attualmente le diverse strutture di ristorazione sono affidate in gestione - in regime di proroga - a ditte diverse, scelte attraverso procedure di gara pubbliche (ristorante dei senatori e mensa del personale) o mediante procedura negoziata (caffetteria del personale e dei senatori). È in corso, peraltro, una procedura di gara europea per l'affidamento in appalto a un solo soggetto della gestione *global service* di tutti i servizi dell'area ristorazione del Senato. del Senato. Il senatore Pedica ha accennato anche alla struttura dei fondi di riserva. Come ha già sottolineato il senatore Comincioli in apertura del dibattito, le previsioni di spesa ipotizzate in via definitiva per l'anno 2009 alla luce anche dei dati conclusivi della gestione 2008 - indicano un fabbisogno finale a crescita zero rispetto al 2008. Abbiamo voluto che lo scenario previsionale del bilancio evidenziasse un più stringente raccordo con i dati della spesa registrata a consuntivo nel 2008, rappresentando una rigorosa espressione dei vincoli contrattuali esistenti, sia per la spesa obbligatoria che per quella di funzionamento, nonché delle decisioni programmatiche e dei conseguenti piani di esecuzione assunti dalla Presidenza e dai senatori Questori. È una decisione che potrà offrire, negli anni a venire, l'opportunità di meglio collegare i dati del consuntivo precedente con la manovra finanziaria del bilancio di previsione. Tale novità ha consentito di offrire oggi una struttura di bilancio previsionale in buona sostanza caratterizzata da una sequenza di saldi negativi sia sulla spesa corrente che su quella in conto capitale. Per converso, è stato assolutamente necessario ipotizzare - comunque nel limite della spesa complessiva a crescita zero, come abbiamo detto - fondi di riserva di consistenza significativa. Nel complesso, siamo di fronte a riserve che crescono - così come è stato sottolineato - di circa quattro volte e mezzo rispetto allo scorso anno, ma sono tuttavia indispensabili in una struttura di bilancio rigorosa come quella disegnata dal bilancio di previsione di quest'anno. Esse, a nostro avviso, non devono apparire eccessive, quanto piuttosto l'espressione di un atteggiamento prudenziale per garantirci un ragionevole spazio di autonomia finanziaria e la possibilità di affrontare situazioni impreviste e nuove decisioni operative con efficacia ed immediatezza. Premesso che è stato avviato un processo di razionalizzazione che riguarda l'assegnazione, la gestione e una più efficiente destinazione degli spazi disponibili, fornisco direttamente le informazioni richieste sulle locazioni. Gli edifici di Santa Maria in Aquiro e Largo Toniolo sono stati affidati dal Senato della Repubblica al Provveditorato alle opere pubbliche al fine di procedere alla loro ristrutturazione edile ed impiantistica. Il Provveditorato gestisce in modo autonomo l'intera procedura, cura la progettazione, affida i lavori e gestisce il cantiere fino all'ultimazione dei lavori, per poi restituire l'edificio ristrutturato. Gli edifici si trovano rispettivamente nelle seguenti condizioni: l'edificio di Santa Maria in Aquiro è stato affidato nel 2003 al Provveditorato che, dopo aver redatto la progettazione e affidato i lavori, li ha dovuti fermare per circa due anni a causa di carenza di fondi. I fondi sono stati reperiti e sono disponibili solo dall'inizio del 2009 per cui solo da allora sono ripresi i lavori. Lo scorso aprile è stata approvata una variante progettuale che ha colmato alcune carenze e ha anche adeguato il progetto sia alle nuove norme nel frattempo emanate che alle nuove esigenze di valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti. La variante progettuale richiede un incremento di spesa ma pare che essa abbia trovato adeguata copertura per cui si spera di attuare il programma che prevede l'ultimazione di circa metà edificio per la fine del 2009 e l'ultimazione di tutti i lavori per marzo 2010. L'edificio di Largo Toniolo è stato affidato al Provveditorato alle opere pubbliche nel 2004. Nella Conferenza di servizi avutasi nel 2005 si è stabilito il cambio di destinazione d'uso ad uffici, necessario al Senato per poter adeguatamente usare l'edificio. La ratifica di tale documento da parte del Comune di Roma si è avuta però solo nel 2008, per cui solo di recente il Provveditorato ha potuto affidare l'appalto congiunto per la redazione del progetto esecutivo e la successiva esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di aprile 2009 e quindi ora il Provveditorato sta avviando l'apertura del cantiere. Il progetto però non è stato ancora inviato al Senato per le valutazioni di rito. In relazione alle questioni sollevate dal senatore Gasbarri, rinvio al parere che il collega Franco esprimerà sugli ordini del giorno, per quanto concerne le concessioni di viaggio a favore dei senatori cessati dal mandato. Quanto alla richiesta di limitare la spesa per i viaggi nazionali dei senatori in carica, esistono due ordini di problemi: in primo luogo, va ricordato che per l'articolo 67 della Costituzione ogni parlamentare rappresenta l'intera Nazione. Egli può quindi esercitare il suo mandato di rappresentante del popolo in qualunque parte del territorio nazionale e non solo nella sede del Parlamento o nel collegio di elezione. In secondo luogo, sarebbe impossibile per gli uffici stabilire volta per volta se il senatore ha viaggiato per ragioni che attengono o meno al mandato parlamentare. L'unico criterio obiettivo sarebbe quello di limitare il rimborso ai soli spostamenti dal luogo di residenza a Roma e viceversa, ma tale disposizione sarebbe in contrasto con le considerazioni che precedono in ordine alla posizione costituzionale dei rappresentanti della Nazione. Quanto alle indicazioni relative al personale, si fa presente che, assumendo i dati i dati relativi alle retribuzioni liquidate del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato (comprensive di ogni indennità e rimborso spese) si è determinato un aumento percentuale del 2,71 per cento tra il 2007 e il 2006 ed invece una riduzione dello 0,15 per cento tra il 2008 e il 2007. Per quanto riguarda invece il costo medio per dipendente di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, si è riscontrato tra il 2006 e il 2007 un aumento del 4,54 per cento e comunque un incremento più contenuto tra il 2008 e il 2007 (più 3,54 Ogni proposta seguirà l'*iter* previsto dal Testo unico (ci riferiamo agli aggiustamenti nelle strutture per snellirle e renderle più efficaci) e pertanto sarà dato tutto lo spazio necessario al confronto e alla trattativa sindacale, argomento richiamato da diversi colleghi. Rispondo con questo anche a quanto comunicato dal senatore Lannutti circa la lettera di CGIL, CISL e UIL. Si terrà conto inoltre per il prossimo bilancio interno delle richieste del senatore Gasbarri circa la previa comunicazione ai senatori di alcuni dati relativi agli organici, al costo medio, alle assenze. Vado rapidamente a concludere. Anche per i prossimi anni, pur nella consapevolezza che stiamo operando su un bilancio a struttura rigida, dove l'86 per cento delle uscite è rappresentato dalla spesa obbligatoria - soltanto il 14 per cento è destinato al funzionamento dell'istituzione, non intendiamo comunque sottrarci ad una sfida che riteniamo doverosa in considerazione della fase particolarmente difficile del Paese. Dopo i tagli apportati con il bilancio di quest'anno, per i prossimi anni sono rimasti ancora pochi margini di manovra, che peraltro intendiamo perseguire con determinazione, in piena sintonia con le direttive del Consiglio di Presidenza. Tutto ciò nella consapevolezza

dei servizi e delle professionalità a supporto del pieno svolgimento del mandato parlamentare. Constatiamo purtroppo con amarezza che finora quasi mai la stampa ha colto il valore di un tale sforzo, essendo invece più attenta a dettagli sulla manovra complessiva, quelli di più scarso rilievo. Non possiamo che auspicare un cambio di direzione in tal senso da parte dei *media*, che sia in grado di porre finalmente l'accento sulle esigenze di funzionalità e di funzionamento dell'istituzione e sul significativo e reale impegno del Senato a razionalizzare, nella massima trasparenza dei dati, la propria spesa riducendo gradualmente il proprio fabbisogno. Ne dà evidenza un bilancio di previsione

collegialmente elaborati dal Collegio dei Questori, e cercherò di farlo in maniera chiara per rispetto ai colleghi che li hanno elaborati ed illustrati, ma anche concisa. infatti opportuno che la chiarezza e la concisione camminino di pari passo. Esprimeremo alcuni pareri favorevoli, di accoglimento, altri

specifico dell'invito al ritiro, nell'eventualità non vi fosse tale assenso, il parere del Collegio dei Questori è da ritenersi contrario. Analizzeremo gli ordini del giorno anche raggruppandoli, perché alcuni spesso toccano, sia pure da un punto di vista diametralmente opposto, lo stesso tema.

gli ordini del giorno G1 e G8 che trattano, in modo però antitetico, la questione relativa al concorso per consiglieri parlamentari, autorizzato dal Consiglio di Presidenza il 16 dicembre 2008. C'è un *excursus* storico da fare

l'indizione del concorso a sette posti di consigliere parlamentare fu approvata dal Consiglio di Presidenza, con le motivazioni - che in altre occasioni, quando si parla di riduzione del personale dipendente del Senato, sono espresse in maniera assolutamente sintetica - così

in particolare: alla sollecita ripresa dei tavoli di contrattazione con le organizzazioni sindacali; all'invio ai sindacati di una documentazione circa i contrattisti a tempo determinato; alla pubblicità degli atti prodotti dai gruppi di studio interni.

si valuteranno le esigenze di documentazione e insieme la possibilità di utilizzare diversamente il personale in servizio per creare opportune sinergie, nonché concrete prospettive relative ai rapporti tra strutture analoghe del Senato e della Camera dei deputati.

Ceccanti e Vita, esso evidenzia l'esigenza di dare certezza giuridica anche alle utenze telefoniche fisse e mobili che questo ramo del Parlamento mette a disposizione dei senatori rispetto ad eventuali attività di intercettazione,

Casson ed altri, si richiede l'installazione di dispositivi di riconoscimento sui terminalidi voto analoghi a quelli recentemente adottati alla Camera dei deputati.

con il posto fisso abbia portato dei miglioramenti in ordine alla corrispondenza fra senatore votante e la propria scheda, il proprio consenso ed il proprio voto. Non ritenendo quindi di accogliere questo ordine del giorno, invitiamo il senatore Casson a ritirarlo.

argomento che, negli ultimi mesi, è stato oggetto di interesse anche in questa seduta, nella discussione generale e nell'illustrazione degli ordini del giorno. In merito, vogliamo ricordare che il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 21 aprile scorso, ha assunto una deliberazione nella quale sancisce, quanto alla possibilità di accredito presso i Palazzi del Senato dei collaboratori dei parlamentari, alcuni principi direttivi

Tra parentesi, presso la Commissione affari costituzionali, ha avuto anche inizio l'esame delle proposte di legge in materia di tipologia di contratto di lavoro dei collaboratori parlamentari. del senatore Paravia, inoltre, chiede che quote del rimborso ai Gruppi parlamentari per le attività di supporto ai senatori siano destinate specificamente agli oneri connessi al rapporto di lavoro dei collaboratori. L'ordine del giorno G11, di cui è primo firmatario il senatore Mascitelli, chiede che il Collegio dei Questori valuti la possibilità di estendere ai collaboratori dei senatori il regime già previsto per i collaboratori dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei Presidenti di Commissione, ossia il versamento diretto da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica dei compensi Ho ricordato quanto prevedono i due ordini del giorno, però, per le motivazioni che ho addotto poco fa, cioè una decisione recentissima già assunta, alla quale sono seguiti provvedimenti del Collegio dei Questori e del Comitato per la sicurezza, non possiamo ovviamente che invitare i presentatori al ritiro degli ordini del giorno G4 e G11, perché riteniamo, come Collegio dei Questori, di aver già dato

Riprendo l'argomento trattato poco fa, a proposito dell'ordine del giorno precedente. Sempre alla luce di una delibera

che ci vedono in stretto contatto con i colleghi Questori della Camera, perché è evidente che il trattamento degli ex parlamentari deve essere sostanzialmente uguale fra Camera e Senato. che questa parte dell'ordine del giorno abbia già trovato sostanziale accoglimento nelle deliberazioni fin qui assunte o in corso di elaborazione. Solo per questo motivo,

si rammenta che la procedura di gara in corso prevede un listino prezzi, che il futuro affidatario del servizio dovrà applicare, più elevato del 40 per cento, rispetto a quello attualmente adottato. È stata, pertanto, già effettuata una scelta che va nella direzione di ridurre il più possibile la differenza tra il listino applicato presso la caffetteria dei senatori e i correnti prezzi di mercato. Accogliamo quindi come raccomandazione

accolto l'ordine del giorno G13, del senatore Mascitelli ed altri, riguardante l'accesso di soggetti diversamente abili

escluse le Commissioni, il lavoro in Aula sia abbondantemente rappresentato nei servizi informatici, mentre per quanto concerne l'informazione di natura patrimoniale, gli incarichi retribuiti, la pubblicazione di questi dati sul sito Internet richiederebbe un adeguamento della legislazione che attualmente disciplina le prerogative parlamentari.

L'ordine del giorno G17, sempre del senatore Perduca ed altri, relativo alla digitalizzazione degli atti delle legislature pregresse, viene accolto come raccomandazione. È una finalità che non possiamo raggiungere immediatamente, ma che potrà essere in un tempo più lungo raggiunta.

con compiti istruttori e propositivi sulla materia. Il tema è molto interessante ed è assolutamente doveroso cercare di dare il più ampio spazio possibile a tutte le attività parlamentari, non solamente a quelle di Assemblea. L'ordine del giorno viene pertanto accolto come raccomandazione. *(Applausi

del mio parere e sul dibattito che si è svolto mi sembra necessaria. Nella relazione scritta avevo tratteggiato alcune linee del percorso che già il bilancio di quest'anno ha iniziato nella riduzione della spesa complessiva del Senato e dei provvedimenti con cui si realizza questa riduzione; nella mia relazione orale avevo ripreso esattamente quella parte, ritenendo che le linee perseguite dal progetto di bilancio sono quelle che, a mio avviso, appaiono convincenti e che sempre più devono essere percorse. si tratta di provvedimenti di medio o lungo periodo, non occasionali, non derivanti da condizionamenti esterni e tendenti alla individuazione ed alla riduzione delle duplicazioni organizzative, delle aree di sovrapposizione gestionale e degli sprechi, ove essi esistano. Credo che questa sia la direzione giusta. Per indicare alcuni grandi elementi che confermano questa tendenza basta sottolineare un dato che mi sembra eclatante. delle risorse finanziarie per il 2009, per la prima volta, rimane identico a quello del 2008, cioè non aumenta percentualmente. Non solo; ma già da qualche anno*... Signor Presidente, ho qualche difficoltà a

registra un risparmio rispetto alle dotazioni iniziali; ciò naturalmente evidenzia una conduzione che già si è incamminata e continua a incamminarsi sulla strada di un certo rigore. Questo è il dato essenziale, insieme ad una maggiore trasparenza dei documenti di bilancio che viene tranquillamente evidenziata in più parti, sia

è pari a meno di un millesimo delle spese dello Stato. Dunque, dobbiamo tutti renderci conto che se la democrazia ha un costo, questo per il Senato è pari a meno di un millesimo delle spese dello Stato.

al netto degli oneri fiscali e di altri oneri per il pregresso, è poco più del 12 per cento del bilancio del Senato.

Credo che il dato fondamentale sia ricordare che l'espressione più alta della sovranità popolare, signor Presidente, cioè le Camere, e quindi in questo caso il Senato da lei presieduto, ha un costo che ormai è di questo tipo. Penso che,

o il lucidascarpe siano grandezze di ordine economico. Vi prego di riflettere su tale i macroaggregati del Senato sono infinitesimi rispetto ai macroaggregati dello Stato. I frazionali di cui parliamo sono, lo ripeto, dell'ordine delle

Non parlo mai di questi argomenti, ma se fosse necessario potrei confrontare il costo di un senatore con quello di tutti coloro che lo criticano. Vi assicuro che il confronto dovrebbe far ritirare

occorre occuparsi di misure strutturali, che intervengono nel tempo e che non pregiudicano la qualità, perché dobbiamo mantenere

quando si agitano strumentalmente l'uno contro l'altro le polemiche indotte dall'esterno, non si fa il bene di nessuno di noi, perché ciascuno poi le tira contro l'altro e ciò significa un arretramento di quella politica nel senso più alto, alla quale credo tutti noi ci ispiriamo, che è quella del governo degli uomini e delle donne. Credo che ciò meriti sempre il massimo dell'attenzione e della dignità.

la Presidenza, tenuto conto del fatto che gli ordini del giorno sistematicamente contengono proposte plurime nelle parti dispositive avendo preso atto del fatto che i senatori Questori, opportunamente, hanno espresso pareri articolati in relazione alle singole questioni, ritiene di dover procedere alla votazione per parti separate, in quanto si tratta di ordini del giorno che, di per sé, si prestano a tale tipo

in quanto durante la discussione generale avevo rilevato che la stabilizzazione del bilancio del Senato è avvenuta attraverso la riduzione degli emolumenti dei senatori e la riduzione dei contributi ai Gruppi e, in parallelo, a una riduzione della spesa in conto capitale, mentre continua ad aumentare la spesa per il personale dipendente del Senato. dipendente del Senato. Non dico che ci sia ancora molto da spremere per quanto riguarda la spesa corrente per i dipendenti, ma allora

è quello di ridurre il complesso della spesa corrente, compresa quella per il personale dipendente, allora mi chiedevo se nel dispositivo si potesse indicare un qualche programma di sfoltimento del personale dipendente, utilizzando il *turn over* o rivedendo l'articolazione amministrativa del Senato; altrimenti la spesa per il personale continuerà a aumentare e questo è incoerente con quanto scritto in questo ordine del giorno.

dove si sottolinea l'esigenza di assicurare una crescente efficienza degli apparati amministrativi, di elevare la qualità delle prestazioni rese al servizio dell'istituzione parlamentare e di adeguamento degli apparati al servizio di una moderna Assemblea legislativa. un generalizzato programma di prepensionamenti che investa tutte le categorie del personale non si tradurrebbe immediatamente in un contenimento della spesa corrente, né in un pronto miglioramento della qualità della gestione amministrativa. Pertanto, anche ove non risultasse sostenibile sul piano finanziario un programma generale di prepensionamenti, appare comunque necessario dotare in tempi brevi l'amministrazione di strumenti di flessibilità organizzativa, tendenti a rispondere a esigenze di ammodernamento e ringiovanimento. Tali strumenti dovrebbero essere assistiti da rigorosi criteri di verifica e valutazione dei risultati, non disgiunti da soluzioni che sappiano valorizzare le esperienze e le professionalità maturate.

del Valori concordi al riguardo - ritirare gli ordini del giorno che abbiamo presentato per cercare di dare il nostro contributo ad un miglioramento dell'impianto, dell'assetto del bilancio interno del Senato.

con alcuni chiarimenti. È vero che sono un parlamentare di nuova nomina, ma il presidente Azzollini, che è veterano delle aule parlamentari, se ha la pazienza di andare a rileggere i Resoconti stenografi

all'eliminazione di privilegi e di *benefit* furono avanzate indistintamente da diversi parlamentari dell'una e dell'altra coalizione;

del giorno - l'accusa di demagogia, di spinte demagogiche e di facile qualunquismo, poco tempo dopo le elezioni politiche del 2008 il Presidente della Camera dei deputati fece una dichiarazione pubblica nella quale, di fronte alla drammaticità della situazione economica del nostro Paese, era contenuto un appello al Governo e alla sua maggioranze affinché si adoperassero per apportare una drastica riduzione dei costi e dei privilegi della politica.

forse questa dignità, presidente Azzollini, va rammentata al Capo del Governo quando chiede una riduzione del numero dei parlamentari, facendo appello ad una raccolta di firme popolare perché ritiene che i parlamentari siano dei tacchini che non possono festeggiare il Natale. La prego quindi di non fare lezioni sulla dignità del ruolo parlamentare a noi dell'Italia dei Valori!

del giorno G8 non viene accettata la proposta del senatore Questore di accoglierlo come impegno a sottoporre le istanze alla Rappresentanza permanente per i problemi del personale, per cui si mette in votazione.

l'insieme delle votazioni, con le votazioni di senatori assenti che si sono verificate e continui richiami, contestazioni e anche tensioni all'interno dell'Aula. Pertanto, l'ordine del giorno in esame mira a impegnare il Collegio dei Questori a promuovere la realizzazione di un impianto di voto sul modello di quello che è stato adottato alla Camera dei deputati, deputati, in modo tale da impedire il voto per gli assenti, peraltro con l'opportunità e con la garanzia delle cautele adeguate ai fini della protezione dei dati personali. Chiediamo la votazione

dei senatori. Troppe volte abbiamo assistito in quest'Aula a scene che francamente non avremmo mai voluto vedere, nonostante l'impegno della Presidenza del Senato. Gradiremmo fare una scelta radicale nell'interesse della credibilità dei senatori.

Francamente, pur apprezzando il lavoro svolto dai senatori Questori e pur condividendo l'impostazione della circolare che pochi giorni fa abbiamo ricevuto (ne ho compreso bene lo spirito), non credo che l'ordine del giorno G4, da me presentato, vada in direzione diversa. Esso pone la questione della soluzione di un problema. La circolare, dal mio punto di vista, lo affronta in buona parte, ma non totalmente; il problema rimane. Bisogna regolamentare contrattualmente questo rapporto di lavoro.

quando il Parlamento aveva in scarsa attenzione il problema del debito pubblico e sono stati concessi perché si riteneva di poterlo fare. A mio avviso, avere oggi appartamenti ad uso abitativo, uffici di rappresentanza e personale per una serie di categorie che ho citato - senatori a vita, ex Presidenti e quant'altro - è eccessivo. Questo costituisce anche un motivo di critica. Io sono lontanissimo dalla demagogia,

un periodo che dà per approvato dalla Commissione un organismo terzo, una sorta di autorità autonoma sulla trasparenza dei conti pubblici. Si tratta di una delle proposte effettivamente avanzate in sede di Commissione bilancio

desidero ringraziare il senatore Morando perché la sua riflessione è corretta, quindi chiedo al proponente di espungere

Signor Presidente, signori Questori, desidero innanzi tutto esprimere, a nome del Gruppo parlamentare UDC, SVP e Autonomie, un sentito apprezzamento ai senatori Questori per il difficile e

Chi vuole parlare cortesemente lo faccia fuori

UDC, SVP e Autonomie, un sentito apprezzamento ai senatori Questori per il difficile e impegnativo lavoro che stanno svolgendo, in particolare per l'impegno per una gestione basata su una politica di controllo e contenimento della spesa, in una situazione con accresciute esigenze di tempestività nel lavoro parlamentare... I nostri ringraziamenti e riconoscimenti vanno a tutta l'amministrazione del Senato, dalla Presidenza e dal collegio dei Questori a tutto il personale, i funzionari ed i collaboratori. Nell'ambito degli obiettivi del progetto di bilancio, mi soffermerò brevemente su alcuni, a mio avviso molto significativi, come per esempio il risparmio energetico. Condividiamo pienamente le scelte e la strada intrapresa dai senatori Questori per migliorare e intensificare l'attenzione al risparmio energetico. L'accordo del Senato con il gestore dei servizi elettrici finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico permetterà non solo un miglioramento dell'efficienza energetica nei nostri palazzi, ma potrà contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e consentire al contempo un risparmio considerevole della spesa sull'energia. La politica del personale sicuramente sarà la sfida più importante per i prossimi anni. Siamo in una situazione Siamo in una situazione di continua crescita di questa posta di bilancio; riuscire a trovare l'equilibrio tra professionalità, ottimizzazione dei servizi e contenimento della spesa richiede un'attenta e delicata gestione e sicuramente una una revisione generale dell'organigramma. Si deve tener conto in questa revisione che la continua evoluzione della telematizzazione e l'utilizzazione del *global service* hanno cambiato in modo sostanziale il lavoro di alcuni servizi dell'amministrazione; ne consegue che il personale dei servizi interessati ha trasformato il proprio lavoro da operativo a lavoro di controllo, di coordinamento e di organizzazione generale. revisione, pertanto, della pianta organica dovrebbe tener conto di queste situazioni per impegnare in modo più razionale le professionalità delle quali ci possiamo vantare in Senato. inoltre, in tutte le decisioni tener presente la programmata riforma del Senato in senso federale. federale. Vorrei soffermarmi inoltre brevemente sull'utilizzo delle sinergie tra Camera e Senato. La scelta della Presidenza e del Collegio dei Questori di continuare con gli interventi volti a un maggior coordinamento ed integrazione dei vari servizi di studio,

il doppio impiego di personale e ottenere un notevole risparmio economico-finanziario. Concludo ribadendo il ringraziamento ai senatori Questori per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo e esprimo anche per conto del mio Gruppo parlamentare il voto favorevole.

nelle precedenti legislature il dibattito sul bilancio interno del Senato è stato animato da diverse valutazioni circa il metodo da preferire nella stesura del bilancio stesso: cassa avrebbe offerto in sostanza una fotografia della contabilità esistente, se al contrario di competenza avrebbe permesso di meglio pianificare e organizzare le questioni di spesa, dando un'indicazione di prospettiva degli impegni assunti. L'annosa questione, poiché una consulenza non si nega mai a nessuno, è stata anche oggetto di un attento studio del gruppo Puoti, Longobardi e Associati che hanno concluso - bontà loro - che l'attuale modello di bilancio offre una lettura più agevole e trasparente della spesa e della gestione. Con tutto il rispetto per gli esperti in materia di contabilità pubblica e soprattutto per il lavoro dei senatori Questori, noi dell'Italia dei Valori vogliamo indicare alcune considerazioni e motivazioni che ci spingono a prendere le distanze da uno sbrigativo atteggiamento di soddisfazione sul bilancio interno della nostra istituzione e vogliamo esprimere le nostre valutazioni sul fragile equilibrio tra la necessità di un reale rigore economico e di un'effettiva trasparenza e, al tempo stesso, il dovere di garantire ai componenti di questa Assemblea le giuste prerogative e non già i privilegi, presentando una diversa chiave di lettura del documento di bilancio che esamineremo da due ottiche o angolazioni diverse: il Senato come istituzione e il Senato come azienda. La prima impostazione è di costante attualità perché investe i problemi della riforma della politica, della credibilità stessa delle istituzioni, del rapporto tra noi e i cittadini. Tutto questo ha tanto più peso e valenza in quanto sappiamo che solo le autonome determinazioni degli organi costituzionali possono decidere la misura del loro concorso

complete, plurali e partecipate delle proprie attività. Non dico questo perché il nostro Gruppo parlamentare, quarto partito in quest'Aula del Senato e in Italia, è stato escluso - forse unico caso in Europa dalla partecipazione alle funzioni e alle competenze e prerogative del Consiglio di Presidenza, mortificando non già la rappresentanza di una singola componente parlamentare, bensì la funzione stessa del nostro Parlamento; perché, a guardare i tempi stretti della disponibilità di esame del bilancio e, in termini di appalti - come diceva stamattina il senatore Pedica - il ricorso non sempre adeguatamente motivato alla trattativa privata, verrebbe da pensare, parafrasando l'espressione di un nostro prestigioso e storico collega, che a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca. Dico questo perché, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, dobbiamo dire che i cittadini non hanno un giudizio entusiasta di tutto ciò che riguarda il lavoro delle istituzioni parlamentari. Sarebbe più che mai necessario un loro più diretto e concreto coinvolgimento, attivando un effettivo ed efficace servizio di informazione a supporto delle attività delle Commissioni, dei singoli parlamentari, della loro attività ispettiva. Sebbene sia stato previsto un aumento del capitolo comunicazione istituzionale, da 10.500.000 euro e 10.900.000 euro, abbiamo trovato del tutto insufficiente che nel documento delle linee guida si parli di un semplice ed ulteriore adeguamento del sito Internet del Senato. poi quanto mai generico il capitolo relativo agli impegni contrattuali per ulteriori servizi televisivi in ordine alla convenzione RAI e al contratto *web* TV. Avremmo poi apprezzato un più incisivo riequilibrio delle risorse messe a disposizione di quelle specifiche attività della nostra istituzione

In un processo di modernizzazione e di democrazia partecipativa, di un confronto vero e non fittizio, i Parlamenti vivono non solo nelle Aule ma anche nelle Commissioni che, per i loro compiti conoscitivi e di indirizzo, devono aprirsi sempre di più alle espressioni della società civile. onorevoli colleghi, aumenta la previsione di spesa delle consulenze, senza alcun intervento di razionalizzazione e di indicazioni normative regolanti la materia. Aumenta il trattamento del personale non dipendente, con importi allineati alla spesa storica del 2008 che tolgono risorse - e lo hanno ricordato anche i sindacati - a quel percorso di formazione e di qualificazione richiesto dall'organico interno. Diminuiscono, invece, le spese connesse alle attività delle Commissioni permanenti, il cui importo complessivo per le attività di indagine è ridotto del 25 per cento. Passiamo ora alla seconda chiave di lettura: il Senato come azienda. Mi rivolgo con particolare con particolare attenzione al senatore Malan nel dire che, come noi tutti sappiamo, in un quadro di organizzazione aziendale di efficienza, è di scarsa utilità prendere come riferimento la spesa storica e considerare se si è speso di più o di meno rispetto agli anni precedenti. Quello che si sarebbe dovuto chiarire nelle Linee guida dell'azione amministrativa è l'indicazione di cosa serva realmente per ottenere quanto si deve fare. che i raffronti tra le poste di bilancio avrebbero dovuto essere presentate con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente piuttosto che agli stanziamenti di preventivo. In questo modo, infatti, si sarebbe ottenuta una percezione più immediata del *trend* di spesa; tralasciamo di dire che l'avanzo di amministrazione avrebbe dovuto essere impiegato per ridurre di pari importo la dotazione ordinaria, proprio in quello spirito di contenimento della spesa pubblica di cui si parla più volte nel documento di bilancio; tralasciamo di dire che l'impinguamento rilevante dei fondi di riserva penalizza una maggiore trasparenza, perché viene meno un'analitica indicazione dei criteri che determineranno le scelte di spesa futura. Ci limitiamo ad alcune considerazioni su alcuni aspetti non marginali del bilancio: sulle spese del personale, dopo avere superato l'annosa questione se la riduzione debba riguardare la pianta organica reale o quella sulla carta, ad oggi non viene ancora proposto ed affrontato in prospettiva un processo di razionalizzazione. Anche questo lo affermano i sindacati interni al Senato. Mille dipendenti sono veramente tanti se comparati con i numeri legali degli altri Paesi. In Inghilterra il personale alle dipendenze della regina non arriva a 800 persone. Da noi, tra costi diretti e indiretti, il costo del personale arriva a 243.818.000, il 41 percento della spesa totale: un costo per addetto che nessuna azienda o impresa di qualunque livello potrebbe sopportare, con un aumento del trattamento stipendiario superiore al tasso di inflazione programmatica, in netta controtendenza con quanto sta avvenendo nel resto del nostro Paese. Sulle spese di rappresentanza questo per evitare demagogia o qualunquismi - è giurisprudenza costante che l'idoneità dell'attività di rappresentanza è quella rivolta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione, dimostrando il nesso temporale o modale tra la spesa e le circostanze che l'hanno originata. Non credo che il Senato sia in sintonia con questi princìpi di buona amministrazione che valgono per tutti. E basterebbe guardare i dati sui servizi dei trasporti: quante auto blu sono attualmente in servizio, quanti contratti di noleggio sono attualmente in vigore? Sugli assegni vitalizi, per sgombrare il campo dall'accusa di facili demagogie, per metterci la coscienza a posto con i cittadini, abbiamo più volte detto - e non solo in questa legislatura, ma anche in quelle precedenti - che gli assegni vitalizi non sono tecnicamente delle pensioni. Va bene che le aliquote contributive sono decisamente più basse in rapporto alla prestazione; va bene che adottiamo un regime di cumulo decisamente più favorevole con altre indennità e vitalizi; va bene che il regime di reversibilità a favore del soggetto superstite avviene indifferentemente dal livello di reddito; va bene tutto questo, ma i primi ad accorgersi che i vitalizi non sono pensioni sono i nostri stessi cittadini perché non vi è nessuna categoria nel nostro Paese che per tempi di maturazione e ammontare delle indennità usufruisce di questo regime di trattamento che, a ragione, viene sentito e percepito come un privilegio. Per queste ragioni, signor Presidente, noi dell'Italia dei Valori voteremo no a questo bilancio perché abbiamo troppo rispetto per il nostro Paese, che in questi ultimi tempi ha raggiunto il triste primato nella classifica OCSE del sesto posto per la più alta disuguaglianza sociale. Voteremo no perché abbiamo troppo rispetto per il Parlamento, che sa bene che rigore economico e morale non possono essere uno slogan, una parola o una formula politica da applicare solo agli altri.

Presidente, il Gruppo del Partito Democratico esprime sostegno al lavoro svolto dal Collegio dei senatori Questori ai quali va dato atto del sostanziale perseguimento di un obiettivo coerente con la permanente riqualificazione della spesa. Va altresì apprezzata l'ampia documentazione a corredo degli atti di bilancio al nostro esame, molto analitici e puntuali. Di assoluto rilievo il minore trasferimento al Senato di risorse finanziarie statali, grazie alle maggiori entrate previste in ragione del contributo aggiuntivo di carattere previdenziale a carico di senatori ed ex senatori per il riscatto del triennio di completamento della XV legislatura, al quale si aggiungono anche 1.800.000 euro di entrate ulteriori determinate dall'incremento dei contributi previdenziali, pagati dal personale dipendente, che sono aumentati dall'8,8 per cento al 9,7 per cento delle loro retribuzioni. Dal lato delle uscite, è degna di rilievo la riduzione delle spese obbligatorie che, come noto, costituiscono la parte più significativa della spesa. Signor Presidente, senatori Questori, anche nel dibattito sul bilancio interno di quest'anno sono affiorate preoccupazioni e sensibilità diverse, nel loro insieme riconducibili al tema dei cosiddetti costi della politica. Già lo scorso anno - anche a seguito delle osservazioni tecniche formulate dal presidente Baldassarri e dal senatore questore Comincioli - fu chiaro come l'esame critico delle situazioni a più riprese denunciate dalla stampa non riguardasse il Parlamento, se non in misura pressoché infinitesimale, come emerso anche nel dibattito odierno e nella replica del senatore relatore. In quella occasione avemmo già modo di sottolineare come la polemica pubblicistica non fosse certamente priva di ragioni sostanziali, specie se riferita alle infinite proliferazioni oggettivamente parassitarie che il sistema politico nel suo complesso ha prodotto negli ultimi decenni. Eppure, signor Presidente, la polemica sui costi della politica in qualche caso ha sconfinato su terreni qualunquistici e sostanzialmente antidemocratici. Va, dunque, riconosciuto agli organi ed agli uffici del Senato - ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza - di aver assunto iniziative volte a ricondurre la situazione nell'alveo del comune sentire di un'opinione pubblica alquanto disorientata e giustamente critica. Di fronte al Paese abbiamo però il dovere di fornire un quadro di elementi certi e trasparenti, rifuggendo in primo luogo da toni vagamente allusivi e ai limiti del vilipendio, allorché, signor Presidente, si lascia intendere senza dimostrazione di alcun elemento oggettivo a sostegno di tesi asserite nel corso del dibattito - che tutta la materia afferente alle gare e ai contratti del Senato sia avvolta in una nebulosa non meglio identificata nei suoi elementi costitutivi. È invece estremamente apprezzabile che il Senato confermi la scelta di una linea di trasparenza, che si esprime attraverso l'affidamento degli appalti con il ricorso a gare pubbliche mediante la piena ed integrale applicazione del codice degli appalti e della normativa comunitaria. Un altro elemento sul quale vogliamo recare un contributo di chiarezza, nel contempo fornendo un indirizzo che ci auguriamo venga coerentemente seguito dal Senato, riguarda le spese obbligatorie in materia retributiva. In proposito, innanzi tutto una precisazione, superflua per gli esperti della materia, ma obbligatoria per i non esperti. Già da tempo la Commissione tecnica per la spesa pubblica, dall'alto del Ministero dell'economia e delle finanze, aveva spiegato l'errore concettuale di collegare la dinamica retributiva al tasso d'inflazione programmata. In quest'Aula, anche nel dibattito odierno, quell'errore è stato ribadito sia pure in modo più sfumato. Per quanto riguarda le retribuzioni parlamentari, è stato detto e chiarito a sufficienza circa i correttivi da intraprendere, ma, ci perdoni, signor Presidente, non potremo mai accettare di sottoscrivere affermazioni udite in quest'Aula di un'indennità quantitativamente scarsa, affermazioni che gridano vendetta, al cospetto di tanti italiani che non riescono ad arrivare alla fine del mese a differenza di noi e dei deputati. È opportuno invece, signor Presidente, sottolineare la proposta che da tempo abbiamo rivolto al Governo di intervenire nelle forme e con le modalità ritenute più opportune al fine di aumentare del 2 per cento l'aliquota sui redditi più alti, fra cui risultano ovviamente quelli dei parlamentari, per destinare queste maggiori entrate alla costituzione di un apposito fondo destinato a tutte le forme di povertà esistenti nel nostro Paese. Per quanto concerne invece le retribuzioni dei dipendenti non è pensabile di ottenere significative riduzioni di spesa, in un'ottica di medio e lungo periodo, se non si procede a riforme di carattere strutturale e permanente. Stupisce in proposito come il lavoro svolto appena un anno fa dalla Rappresentanza permanente del Consiglio di Presidenza per i problemi del personale e rassegnato nelle mani del Presidente del Senato, con nota del 29 febbraio 2008, non abbia avuto seguito alcuno. In quel documento veniva prevista, accanto all'introduzione del sistema contributivo per i nuovi assunti, una maggiore flessibilità operativa dei dipendenti e una riduzione complessiva delle figure professionali di carattere meramente esecutivo, invertendo quindi l'attuale dinamica della progressione economica delle carriere, in coerenza con la maggiore permanenza in servizio garantita per il futuro. Solo in tal modo, signor Presidente, si potrà garantire l'elevata qualificazione professionale tradizionalmente garantita dall'amministrazione del Senato e procedere ad ulteriori economie gestionali; ogni altro strumento rischia di risultare soltanto demagogico e controproducente. I risparmi di spesa sono ora cospicui ed evidenti e di questo va positivamente dato atto sia al Collegio sia all'Amministrazione; non sarebbe pensabile, però, garantire efficienza e tempestività ove ad essi fossero continuamente rivolte richieste indiscriminate e non ragionate di riduzioni di ogni ordine e grado. Al riguardo, nel dibattito della seduta antimeridiana è stato opportunamente sottolineato come lo sbarramento posto nei concorsi per consiglieri parlamentari del Senato effettuati negli ultimi anni con il ricorso al voto massimo di laurea quale requisito per l'ammissibilità alle prove scritte, sia solo apparentemente più garantista in quanto, in realtà, favorisce i laureati di quelle università che producono scarsa qualità a fronte di altissime votazioni concesse per garantire la sopravvivenza di corsi e docenti non adeguatamente competitivi. L'osservazione per la quale un «bocconiano» non partecipa ai concorsi del Senato perché ritenuto inadeguato se laureato con una votazione inferiore al massimo, spiega tutta l'insufficienza di una scelta che va rivista in direzione delle modalità tradizionalmente garantite da altri organi costituzionali, che selezionano il meglio e a costi di gestione dei concorsi più contenuti. Signor Presidente, altre misure sollecitate da colleghi possono trovare adeguate soluzioni in una programmazione pluriennale degli interventi, che dovrebbe essere introdotta anche al fine di un esame comparativo dei bilanci di cassa, attualmente in essere, e delle rispettive voci di competenza. È necessario continuare ad incoraggiare la permanente razionalizzazione della spesa, rifuggendo al contempo dal rischio di assecondare una critica ed improduttiva negazione del ruolo centrale che l'Istituzione parlamentare ha per la vita democratica del nostro Paese.

al suo magistrale intervento a sostegno della sua già nitida relazione, che ha svelato un punto di vista che appartiene a tutti,

Infatti, è forse la seconda volta che il Senato riesce a valutare il rendiconto dell'esercizio precedente in quello immediatamente successivo, anche se con lieve ritardo sul previsto dovuto al calendario parlamentare. Ciò consente di fondare su basi sempre più certe le previsioni per il 2009 e per il biennio successivo. Le entrate del 2008, pari a poco più di 600 milioni di euro, danno una sostanziale conferma delle previsioni iniziali e mostrano un aumento di oltre il 3 per cento sul dato definitivo del 2007. Le spese complessive (oltre 532 milioni di euro) fanno registrare una riduzione significativa rispetto al dato iniziale (594 milioni), e un aumento di poco più del 2 per cento rispetto al dato finale del 2007. del 2007. Tale dato indica l'incremento della spesa, ma all'interno delle decisioni assunte dal Consiglio di Presidenza per l'esercizio scorso di fissare un tasso di crescita della spesa non superiore al 2,5 per cento. Ricordo che la decisione in questione prevedeva che il tasso di crescita della spesa fosse non superiore a quello del PIL nominale fissato dal DPEF del triennio 2008-2010. Le previsioni per il 2009 vedono le entrate e le spese complessive fissate in poco più di 594 milioni di euro, come ricordava così bene il presidente Azzollini prima, riproponendo il dato previsionale del 2008. Le entrate, che nelle previsioni del 2008 erano in aumento significativo rispetto all'anno ancora precedente, dimostrano una riduzione rispetto al dato consuntivo, che era di 600 milioni di euro, data da una crescita molto contenuta della dotazione ordinaria (cioè la posta essenziale per il funzionamento dell'Istituzione) e una riduzione significativa del fondo cassa iniziale (oltre il 20 per cento). Invece, le spese nei primi due titoli, considerate al netto dei fondi di riserva, evidenziano un incremento inferiore all'1 per cento rispetto al dato consuntivo del 2008 e, addirittura, una contrazione di oltre il 2 per cento rispetto al dato previsionale del 2008. Tutto ciò a dimostrazione di una chiara volontà di perseguire obiettivi concreti di contenimento e razionalizzazione della spesa. che la previsione della spesa del Senato nel quadro comparativo della spesa complessiva dello Stato costituisce, come meglio è stato fatto notare da altri relatori prima, lo 0,079 in calo rispetto, ad esempio, all'anno finanziario 2007, che, nel quadro più complessivo della spesa dello Stato, dello 0,085 per cento. In quell'anno la maggioranza era di tutt'altro segno. È evidente che è sembrata a tutti opportuna, ma soprattutto oculata, la scelta di non attribuire al solo bilancio 2009 l'avanzo di esercizio 2008 (pari ad oltre 67 milioni di euro), ma di spalmarlo sugli esercizi successivi, in vista di progressive riduzioni di tale posta, dovute alle modificate dinamiche delle entrate

la riflessione sull'adozione di una diversa metodologia di costruzione del bilancio interno, documento che consente di «leggere» l'Istituzione, dovuta forse, non solo all'aggravio economico ed organizzativo che avrebbe comportato (soprattutto in questo momento), ma anche alle disposizioni in materia di redazione dei bilanci pubblici contenute nella riforma della contabilità pubblica, in corso di esame ed approvazione proprio in queste ore in quest'Aula; l'intercameralità di alcuni servizi, peraltro resa definitiva in alcuni casi come il Servizio bilancio previsto nella citata riforma, che certamente verrà strutturata in modo da non ledere l'autonomia di entrambe le Camere sancita costituzionalmente; la rivisitazione delle spese per gli investimenti (quelle in conto capitale). Dicevo prima che margini di miglioramento si intravedono nella gestione delle risorse per il personale dipendente e questo sta a cuore a tutti. Giusta è la direzione intrapresa dalla razionalizzazione (la già detta intercameralità, i possibili accorpamenti di funzioni, la riduzione degli sprechi e di quant'altro sia necessario), che comporterà sicuramente recuperi significativi di efficienza: un miglioramento quantitativo essenziale che, però, non può e non deve andare a detrimento della qualità e dell'eccellenza raggiunta da questa Istituzione. Anche sulla qualità del servizio fornito si misurano il il risultato e l'ottimizzazione della nostra spesa. È quindi necessaria una politica per il personale, che significa innanzitutto programmazione di piante organiche e di funzioni, non a breve termine; individuazione delle reali necessità operative di una struttura in trasformazione da tempo, ad esempio, che si lamenta l'insufficienza di funzionari per le Commissioni e un ordine del giorno presentato dai Presidenti lo ha evidenziato); previsione di percorsi di inserimento, di carriera e di incentivazione di professionalità adeguate, evitando di incorrere nell'equivoco, spesso coltivato (talvolta anche in questa Aula), che è il numero a fare la forza delle Istituzioni. È invece la qualità a fare la forza di un servizio pubblico in generale, e in particolare di quello di cui oggi parliamo. A me pare particolarmente apprezzabile, tra le tante cose che potremmo mettere in evidenza, l'aver condotto con equità e lungimiranza, nell'ambito dell'accordo con le organizzazioni sindacali del personale dipendente, da parte della vice presidente Rosi Mauro, su delega del presidente Schifani e dell'intero Consiglio di Presidenza, la riforma degli incentivi economici, al fine di evitare la corresponsione generalizzata e indifferenziata di indennità non commisurate ad un effettivo miglioramento della produttività e ad un concreto incremento di efficienza; tutto ciò in linea con i più recenti indirizzi di riforma del lavoro pubblico. Questo ha determinato non solo uno di quei risparmi che hanno consentito al Senato Grazie, di una totale aderenza della gestione amministrativa e politica alle migliori strategie di riforme per la modernità e la trasparenza. Sono certa, peraltro, che in questo sforzo di innovazione nella ricerca e nell'attuazione di politiche più incisive ed innovative l'amministrazione del Senato saprà, come è nella sua tradizione, svolgere un ruolo determinante. A questa amministrazione indispensabile supporto dell'istituzione parlamentare per lo svolgimento del nostro mandato, della Presidenza, dei singoli senatori desidero in questa sede manifestare il più vivo apprezzamento e annunciare il voto favorevole al bilancio del Senato da parte del Popolo della Libertà.

a conclusione del dibattito, voglio ringraziare tutti coloro che sono oggi intervenuti. In primo luogo, il ringraziamento va ai colleghi senatori Questori, al presidente Azzollini e a tutti i Presidenti di Commissione, che hanno dato il loro contributo, unitamente ai membri del Consiglio di Presidenza, per la definizione dei nostri documenti contabili. Per quanto riguarda il Consiglio di Presidenza, voglio di nuovo invitare i Gruppi parlamentari a trovare una soluzione concordata ed equilibrata che garantisca a tutti i Gruppi una loro legittima presenza in quell'organismo. Ho seguito con attenzione gli interventi svolti, pur se impegnato in appuntamenti istituzionali in buona parte della giornata. Tutti coloro che sono intervenuti, anche quelli che lo hanno fatto in maniera, a volte, fortemente critica, hanno contribuito ad arricchire il dibattito con osservazioni e proposte che meritano una riflessione ed una risposta. I colleghi Questori in sede di replica e di esame degli ordini del giorno hanno già fornito le loro risposte, ma ritengo che sia necessaria una riflessione ulteriore che dobbiamo senz'altro a voi senatori, ma in primo luogo all'opinione pubblica. In tutti gli interventi, anche in quelli più critici, ho tuttavia potuto cogliere il riconoscimento di un percorso che, per alcuni in modo ancora non completamente soddisfacente, è già avviato. Un percorso che risponde ad esigenze diverse, sulle quali è assai attenta la pubblica opinione. In primo luogo, quella di una utilizzazione prudente e ottimale delle risorse che lo Stato, in particolare in un momento delicato come questo, mette a nostra disposizione. In secondo luogo, la necessità che il Senato non solo appaia, ma sia realmente una casa di vetro per i cittadini. Ancora, che quanto viene speso venga speso bene, per un corretto ed efficiente funzionamento dell'istituzione parlamentare. Il Parlamento è il bene primario della nostra democrazia; ad esso, anche nei momenti di critica più dura, guardano sempre i nostri elettori. La critica, anche severa, a noi parlamentari non deve mai essere rivolta all'istituzione che rappresenta milioni di cittadini. Ma anche la critica ai parlamentari non deve mai ignorare l'impegno, la competenza, a volte il vero e proprio sacrificio che tanti di voi quotidianamente e in silenzio dedicano al proprio lavoro. La difesa del Parlamento, la tutela della sua autonomia, il miglioramento della sua funzionalità e delle sue strutture sono un dovere che abbiamo non solo nei riguardi di noi, che nel Parlamento viviamo quotidianamente, ma in primo luogo nei riguardi dei cittadini e dell'intero Paese. Grazie, quindi, di nuovo a tutti voi, a coloro che quotidianamente ci aiutano nel nostro lavoro, ma anche a tutti coloro che, a cominciare dalla stampa, possono con le loro osservazioni, anche critiche, aiutarci a migliorare la nostra attività. *(Applausi

manifestazioni soppresse con la violenza e anche a seguito di quanto auspicato da colleghi della Camera, riteniamo anche noi di unirci alla richiesta rivolta nei confronti del ministro Frattini di riferire alle Camere su qual è l'atteggiamento dell'Italia, adesso che è acquisita la non partecipazione dell'Iran al prossimo G8 di Trieste, che avrebbe dovuto parlare

gravi anche da parte del Consiglio dei chierici iraniani che ritengono che oltre 3 milioni di voti sono in esubero rispetto a quelli che sono stati in effetti conteggiati. È stata da loro manifestata una una disponibilità a fare un riconteggio più approfondito. Io credo che invece la questione vada presa in considerazione nella sua totalità. Chiaramente l'Italia da sola non lo può fare, ma occorre sapere qual è la posizione del ministro Frattini, anche all'interno dell'Unione europea, relativamente alla questione che - ripeto

che lavorano sul totale della popolazione e che si colloca ai primi posti in Europa ed al primo posto in Italia per l'indice di povertà, visto che più del 30 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, voglio esprimere la solidarietà ai lavoratori della FIAT di Termini Imerese e dell'indotto che rischiano il loro posto di lavoro.

visto che la FIAT ha trapiantato in Serbia alcune attività previste per Termini Imerese, come le presse per la produzione della componentistica; responsabilità che hanno annullato 5.000 nuovi posti di lavoro. Ma la dismissione della produzione automobilistica dello stabilimento siciliano è inaccettabile. Non si possono cancellare professionalità che hanno alimentato il prestigio del marchio FIAT producendo i modelli più venduti; e la distanza dai circuiti di commercializzazione pare un alibi che offende l'intera Sicilia e il Mezzogiorno. Imerese c'è il porto e dovrà esserci l'interporto. Si producano autoveicoli utilizzando un *know-how* tecnologico con forte impronta ecologica che sia da apripista per la salvaguardia dell'ambiente con uno spiccato *appeal* per le giovani generazioni. *(Applausi

una parte dei colleghi del Partito Democratico apporre un fiocco verde sui baveri delle giacche e sui vestiti. Abbiamo capito che si tratta di un'azione di solidarietà nei confronti del popolo iraniano, speriamo anche di viva condanna del regime e della repressione che sta attuando e pertanto di solidarietà alle vittime. Noi della Lega amiamo fregiarci spesso, anzi costantemente, di un sigillo verde;

della nostra Aula e del Parlamento. Credo che, al di là di rivendicazioni giuste e di coerenze richieste, noi dovremmo affermare la dignità della nostra Aula esercitando appieno le nostre funzioni.

dalla passata legislatura, in cui c'era il tempo e il modo di fare una riforma su un testo *bipartisan*, a tutto quest'anno, l'Aula non l'ha fatta.

dell'uso del *referendum* e cerca di innovare. So che la risposta che mi verrà dalla Presidenza è di parlarne all'ufficio di Presidenza della Commissione e domani lo farò, ma ho voluto fare questo intervento perché tutta l'Aula ne fosse informata. Poiché il ministro Maroni ha detto che verrà fatta una proposta di legge, voglio informare la Presidenza e tutta l'Aula che si parla di una materia d'iniziativa

Il senatore Divina ha testimoniato la solidarietà anche del Gruppo della Lega Nord al popolo iraniano. Evidentemente non sono solo i senatori del Partito Democratico e della Lega a portare questo nastro o comunque ad essere solidali con il popolo iraniano. Credo che sia una cosa una cosa positiva che questa solidarietà, che ci auguriamo sia operante e trovi risposta, sia condivisa da tutti i Gruppi parlamentari.

cercare di ovviare alle debolezze della legislazione attuale, ma anche di proporre nuove forme di effettiva democrazia diretta per dare al popolo quello che gli spetta, naturalmente il potere di copartecipare alle decisioni importanti della